ordine del giorno: Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti

recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche´ per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo

1. Allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza, anche in ambito comunitario, in relazione alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare,

in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche´ per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (2665) (Relazione

esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.300 e 7.3,

Prego,

nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi di pubblicita, imparzialita, paritadi trattamento, trasparenza e proporzionalita previsti dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163,

sullo stato di realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento ai sensi del comma 4, al fine di verificare l’esatto adempimento delle condizioni e degli obblighi richiesti».